della maggioranza presentato, nei termini, venerdì scorso. Riguarda, in particolare, tutte le questioni relative al regime transitorio, cioè quelle che in questa fase e per questa parte del provvedimento più ci preoccupano,

per le intercettazioni e la pubblicazione degli atti. Ricordo, sinteticamente, quali sono le norme che entrerebbero in vigore subito, se dovesse essere approvato questo disegno di legge. Tali norme riguardano, oltre gli obblighi di astensione del giudice e del pubblico ministero, ministero, le intercettazioni nei confronti del difensore, i divieti di pubblicazione, l'obbligo del segreto (che ora sarebbe esteso anche all'attività, oltre che agli atti di indagine); riguarderebbero, inoltre, il divieto di trascrizione di parti di conversazioni relative a terzi, a terzi, la violazione dell'obbligo di segreto per le intercettazioni, le comunicazioni all'autorità ecclesiastica (in determinati casi, per procedimenti relativi ad ecclesiastici) e le riprese audiovisive del dibattimento.

quello che sarà o potrebbe essere un suo giudizio nelle prossime ore, ho però necessità di ribadire quanto noi abbiamo già chiesto nella

stiamo discutendo un provvedimento importante che, a nostro avviso, imbavaglia l'informazione, anche nella forma

che il testo licenziato dalla Commissione sarebbe stato oggetto di un approfondimento e di un confronto anche con le opposizioni - ritengo io - prima di giungere all'esame dell'Aula. Sulla scorta di questo, peraltro, si era anche lasciato intendere che c'era la possibilità di introdurre elementi di particolare novità sul testo. Già la calendarizzazione rapida di questo provvedimento ci ha creato una serie di problemi. Noi abbiamo appreso dalla stampa, prima, e poi letto che il Gruppo parlamentare del Popolo della Libertà ha presentato una serie di emendamenti

l'ambito di immediatezza dell'operatività della norma transitoria sulla legge delle intercettazioni, che non ci sembra sinceramente un buon viatico.

con le opposizioni e, comunque, rispetto al metodo annunciato vi è stato un altro modo di comportarsi. È nel diritto della maggioranza; forse, se ce lo avessero detto prima, avremmo solo perso qualche giorno in più in Commissione. Il Il tema qual è? La richiesta venuta dai colleghi del Partito Democratico di un rinvio in Commissione del testo, in considerazione anche dei nuovi emendamenti proposti dalla maggioranza, è una questione è una questione che andrebbe esaminata e decisa ora, prima di discutere delle pregiudiziali di costituzionalità in ordine al testo. Altrimenti ci troveremmo con un doppio lavoro che, sinceramente, non capisco dove possa portare: ci pronunceremmo infatti ora sulla costituzionalità o meno del testo e poi, eventualmente, qualora - in un caso su mille - si dovesse pensare di fare un approfondimento in Commissione,

Signor Presidente, noi nel merito non siamo d'accordo. Rinviare tutto il provvedimento in Commissione, com'è stato richiesto dal senatore Belisario e da altri Capigruppo, è una proposta che non possiamo accettare. La Commissione discute di intercettazioni - lo ricordo a quest'Aula - da più di un anno qui al Senato; è giunto dunque il momento, per quanto ci riguarda, di affrontare il tema seriamente in Aula.

questo è un buon testo, che reca una normativa equilibrata, che va a garantire tutti. Garantisce i magistrati, che potranno utilizzare le intercettazioni nelle indagini: tutti i reati che ora sono intercettabili saranno garantiti e confermati, con l'aggiunta dello *stalking*. Garantisce la libertà di stampa, perché al Senato abbiamo trovato

sarà facoltà del Presidente - e noi ne prenderemo atto - svolgere, dopo l'incardinamento, le dovute considerazioni del caso ed eventualmente trovare altre soluzioni. intervengo per offrire due elementi alla sua valutazione.

che ha esposto il presidente Zanda. Vorrei dire solo due cose. Non può essere invocata la necessità di fare presto, nel senso che non può essere invocata *contra* l'opposizione,

a discutere di emendamenti presentati dal relatore di maggioranza e appoggiati dal Governo; dopodiché, la stessa maggioranza e lo stesso Governo ci hanno ripensato e, quindi, tutto quello che abbiamo discusso si è rivelato del tutto inutile. Ma certo non siamo stati noi a "remorare" la discussione e l'approvazione del provvedimento. Per questo trovo bizzarra l'argomentazione adoperata dal presidente Bricolo. La seconda questione è più tecnica, signor Presidente. Poc'anzi, era intervenuta questione in ordine alla sospensione della nostra discussione d'Aula e al rinvio del provvedimento in Commissione e si è fatto riferimento all'articolo 100, comma 11, del Regolamento. In realtà, mi permetto di dire che l'articolo 100, comma 11, del Regolamento prevede un ritorno in Commissione incidentale durante la discussione del provvedimento.

stiamo alludendo anche ad una questione molto più rilevante, più complessa e politicamente, secondo me, più consistente: il fatto cioè che non è possibile che un provvedimento come questo,

e nell'opposizione, su almeno cinque questioni, pare ci sia la possibilità di riaprire una discussione. Presidente, il nostro Gruppo non ritiene necessario un ritorno in Commissione del provvedimento. Discuteremo nel merito nella discussione generale e nel voglio intanto dire che la discussione su questo provvedimento è stata lunga, seria ed approfondita. Il provvedimento fu presentato il 30 giugno 2008, 23 mesi fa.

dal luglio 2008 fino al giugno 2009. Quindi, le sedute che ho citato si sono svolte durante l'arco di un anno, a conferma che si è trattato e si tratta di un provvedimento

abbiamo avuto 38 sedute in Commissione. Non ho qui dati di raffronto, ma credo che sia una trattazione che, difficilmente, possa trovare precedenti di analoga o superiore durata: 38

Più volte il Presidente del Senato in Conferenza dei Capigruppo ha rivolto degli appelli al fine di posticipare di alcune settimane questa discussione. Noi abbiamo accettato gli inviti del Presidente del Senato perché,

Per quanto riguarda gli emendamenti, devo dire che anche in sede di Conferenza dei Caprigruppo - la presidente Finocchiaro lo dovrebbe ricordare - dissi che, se avessimo presentato emendamenti rilevanti, lo avremmo fatto prima dell'esame in Aula,

di emendamenti non meditati, ma di riflessioni che abbiamo svolto anche sulla base del dibattito tenutosi in Commissione e nel Paese. Essi riguardano non solo l'entrata in vigore della legge, ma anche la pubblicazione di materiale proveniente da procedimenti giudiziari e altre vicende che sono notissime e che sono al centro del dibattito.

ho visto che in questi giorni la stampa e le televisioni hanno dedicato molta attenzione a tali emendamenti. Subito li abbiamo pubblicati integralmente sul sito *web* del Gruppo, e ho visto che questa comunicazione è stata ampiamente ripresa dagli addetti ai lavori.

in Commissione: tra l'altro, molti emendamenti ripristinano testi già precedentemente votati dalla Camera dei deputati o in altre fasi della discussione, a conferma del fatto che i dibattiti sono necessari anche per maturare dei convincimenti. Dunque, se ci si blinda e non si cambia nulla si è dalla parte del torto; se si fanno riflessioni e si corregge qualcosa, non va bene: mi pare un po' pretestuosa la posizione delle minoranze, che dovrebbero prendere atto del fatto che abbiamo maturato delle posizioni innovative, che si rifanno anche a fasi di dibattito precedente. Quindi, concludendo, signor Presidente, riteniamo che dopo due anni di intense discussioni nelle Aule e nelle Commissioni si possa procedere. Presidente

quale questa Presidenza si è riservata di pronunziarsi durante l'andamento dei lavori di questo disegno di legge, riserva che si impegna a sciogliere

Il principio è stato introdotto in Commissione e vi è un emendamento che ne amplia la portata. l'immediata applicazione degli articoli 36 e 53 in ragione di un diverso regime dell'articolo 114,

una lunga sequela di norme che modificano il codice di procedura penale, non solo con riferimento alla procedura vera e propria delle autorizzazioni alle intercettazioni telefoniche, alle intercettazioni captative di immagini visive e alle intercettazioni cosiddette ambientali, ma anche ad una serie di norme che ne sono corollario, non solo del codice di procedura penale, ma anche del codice penale ed in altre leggi che andrò elencando. Viene introdotta all'articolo 36 del codice di procedura penale una nuova ipotesi di astensione per dichiarazioni rilasciate dal magistrato affidatario del procedimento, che ha un riferimento nell'articolo 53 dello stesso codice di rito, ai fini della sostituzione del magistrato o del pubblico ministero che si trova ad essere affidatario del procedimento, a causa di queste dichiarazioni, se vi è stata anche, tra l'altro, una denuncia con iscrizione nel registro degli indagati per il reato di cui all'articolo 379-*bis*, cioè rivelazione di segreto da parte del pubblico ufficiale che ne ha avuto conoscenza a causa del proprio ufficio. In tal caso, la sostituzione è possibile

il capo dell'ufficio che decide in base all'articolo 11, cioè nel distretto viciniore, sul procedimento su cui la denuncia è scattata. accentuato il divieto assoluto di intercettazione del difensore anche su un'utenza diversa da quella da lui utilizzata, con una sanzione disciplinare, nel caso di annotazione di informativa anche verbale di tale intercettazione. Viene ad essere esclusa nel testo approvato dalla Commissione - vedremo poi come gli emendamenti presentati dalla maggioranza hanno modificato questo punto punto - la possibilità di pubblicazione di atti di indagine fino alla chiusura delle indagini preliminari e all'udienza preliminare. Viene prevista la pubblicazione solo nel contenuto dell'ordinanza di misura cautelare dopo la conoscenza da parte dell'interessato, fatta eccezione per le parti riguardanti le comunicazioni e i relativi flussi. Al riguardo, vedremo successivamente come anche nell'ordinanza di custodia cautelare il riferimento alle intercettazioni possa essere fatto solo nel contenuto. Viene previsto il divieto di pubblicazione di immagini dei magistrati, a meno di un'impossibilità di separare le immagini dalla cronaca del fatto, così come viene previsto il divieto di pubblicazione delle comunicazioni da distruggere, che sono quelle relative ai terzi estranei

e degli atti relativi ad intercettazioni illegali, vengono aggiunti i documenti e i supporti illegali relativi alle condotte sanzionate dal nuovo articolo 616*-bis* del codice penale introdotto nel disegno di legge in esame, di cui tratterò nel prosieguo.

la ripresa di immagine captativa della conversazione, nel concetto omnicomprensivo di intercettazione, e si prevede poi una distinzione con l'acquisizione della documentazione, e cioè dei cosiddetti tabulati. tabulati. Rimane assolutamente identico al testo vigente l'elenco dei reati intercettabili, tranne che per l'aggiunta del reato di *stalking*, perché tra i vari

Per quanto riguarda le intercettazioni tra presenti - le cosiddette intercettazioni ambientali - esse vengono previste solo nei luoghi ove vi è fondato motivo di ritenere che si stia svolgendo l'attività criminosa.

distinguendo tra quelle captative e quelle semplici, che possono essere svolte anche su iniziativa della polizia giudiziaria senza necessità di autorizzazione da parte del magistrato; il secondo tratta dell'intercettazione di corrispondenza postale. penale si entra nella prima grande innovazione del sistema, perché l'autorizzazione a poter intercettare viene richiesta dal pubblico ministero, naturalmente con l'assenso scritto del procuratore della Repubblica o del procuratore aggiunto o di magistrato delegato,

delle indagini preliminari che ha sede nello stesso ufficio dove svolge la sua attività di pubblico ministero, come nel testo vigente. Devono concorrere congiuntamente i seguenti presupposti: gravi indizi di reato (già esistente nell'attuale testo vigente), indispensabilità alla prosecuzione delle indagini (già esistente nell'attuale testo vigente) con una specificazione ai numeri 2, 3 e 4 che vede il riferimento alle intercettazioni e alle intercettazioni d'immagini). Mi riferisco, cioè, alla necessità che l'utenza da intercettare sia intestata all'indagato, ovvero sia utilizzata abitualmente ed effettivamente da lui (quindi, può essere intestata anche a terza persona), ovvero che si possa intercettare l'utenza di persona comunque a conoscenza dei fatti per cui si procede, vi è motivo di ritenere che le conversazioni verteranno sui fatti per cui si procede (peraltro, tale circostanza anche oggi, ancorché manchi nel tessuto normativo, dovrebbe comunque essere valutata dal magistrato per poter indirizzare su alcuni soggetti ben precisi). Viene prevista la trasmissione di tutti gli atti d'indagine al tribunale e, ai fini della valutazione della gravità dei fatti, vengono richiamati gli articoli 192, commi 3 e 4 commi 3 e 4 (valutazione delle dichiarazioni di imputati in procedimenti connessi o collegati, che va fatta insieme ad altri elementi presenti nell'indagine), 195, comma 7 (valutazione della testimonianza di chi non vuole rivelare la fonte da cui proviene la notizia), e 203 (dichiarazione derivante dal cosiddetto informatore)

la durata viene fissata in 30 giorni, prorogabile di altri 15 giorni *sic et simpliciter*, con un'ulteriore proroga di altri 15 giorni nel caso continuino a ricorrere i presupposti e, ove vi siano nuovi elementi che emergono dalla intercettazione, con un'ulteriore un'ulteriore proroga; pertanto, si arriva complessivamente a 75 giorni per impedire ulteriori conseguenze all'attività criminosa o la commissione di nuovi reati.

organizzazioni criminali che però non sono considerate di stampo mafioso), la durata delle intercettazioni rimane assolutamente identica:

Rimane il presupposto di partenza, cioè i sufficienti indizi di reato, esattamente come oggi; quindi, in buona sostanza, per questo tipo di reati la normativa non viene modificata. Lo stesso vale per le intercettazioni cosiddette ambientali, che non vedono alcuna novità al riguardo. viene previsto un apposito registro nel quale devono essere annotati i dati del decreto, il momento in cui comincia la disciplina delle operazioni d'intercettazione, il verbale; i supporti devono essere conservati in archivio riservato; vengono attribuiti al procuratore generale e al procuratore della Repubblica poteri di controllo, vigilanza e gestione dei centri di intercettazione; al termine delle operazioni si prevede la trasmissione dei verbali al pubblico ministero,

anche per evitare *discovery* anticipate per reati di altro tipo per i quali non si sta procedendo e che potrebbero essere emersi casualmente nel corso delle intercettazioni. Viene dato agli avvocati un termine non inferiore a 15 giorni per l'esame, che può anche essere integrale, nel senso che si può ascoltare l'intera registrazione. È prevista un'autorizzazione per ragioni di indagine da parte del tribunale ad un ritardato deposito. Viene prevista un'udienza stralcio,

fatti personali e, quindi, una materia che deve rimanere estranea al procedimento in quanto assolutamente irrilevante, con alcuna conseguenza su di esso. tali parti viene enunciato il divieto di trascrizione. L'articolo 269 del codice di procedura penale prevede l'archivio riservato per i verbali e i supporti e la loro distruzione comunque dopo il passaggio in giudicato della sentenza per il fatto per cui si procede.

(procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato), 257 (spionaggio politico o militare), 416-*ter* (scambio di voti con organizzazioni mafiose),

il caso in cui viene richiesta l'autorizzazione ad intercettare un'utenza che si sa appartenere ad un soggetto che lavora per i servizi di sicurezza: si prevede allora che il procuratore della Repubblica

del reato per il quale la legge non prevede l'autorizzazione dell'intercettazione; spesso molti reati vengono iper-rubricati proprio per ottenere strumenti investigativi che in realtà la legge non prevede. D'altra parte, se essi fossero rubricati correttamente, non si arriverebbe all'intercettazione.

Tizio e Caio parlano di questo e da ciò deriva la circostanza che Tizio è autore del reato e svolge un certo ruolo nell'ambito del fatto per cui si procede. All'articolo 293 si prevede la facoltà dell'esame integrale dell'intercettazione da parte del difensore, con riferimento all'ordinanza di custodia cautelare che, vedendo un richiamo solo nel contenuto, limita *prima facie* la possibilità di difesa e quindi la necessità da parte del difensore di prendere cognizione integrale dell'atto. di procedura penale prevede l'autorizzazione alla pubblicazione di singoli atti o di parti di intercettazioni utili alle indagini, con una anticipazione della pubblicità utile al riguardo.

269, accennato in precedenza, e sui dati acquisiti illecitamente fino alla chiusura delle indagini preliminari. di attuazione che fissano i funzionari amministrativi di polizia giudiziaria e di cancelleria responsabili della tenuta dei registri e dell'archivio riservato.

rappresentante della Chiesa, già esistente nell'attuale nostro ordinamento, la quale però viene specificata con riferimento al grado ricoperto nell'ambito della gerarchia ecclesiastica. Infine, all'articolo 380, comma un ampliamento dell'arresto obbligatorio in flagranza di reato anche per il furto aggravato commesso nell'ambito di una associazione a delinquere, nonché per gli atti sessuali

L'articolo 614 del codice penale viene ampliato nel raggio di azione. Parliamo della cosiddetta violazione di domicilio, cosiddetta violazione di domicilio, dove il concetto di privata dimora viene sostituito da luogo privato. Si tratta, quindi, di ampliamento complessivo. Alcune di queste norme erano collegate

maggioranza - professionisti iscritti all'albo professionale nell'esercizio del diritto di cronaca. Esiste, però, già un ampliamento contenuto in alcuni emendamenti. Vi è poi un adeguamento alle nuove norme dell'articolo 617

individuate le sanzioni per gli editori in caso di pubblicazione di notizie coperte da segreto, con la previsione della pena da 250 a 300 quote.Vi è una procedura di rettifica che riguarda i siti informatici, ivi compresi quotidiani e periodici diffusi in rete senza commenti. Si ipotizza una procedura che per quanto riguarda il profilo economico...

ci sono norme che riguardano gli stanziamenti e le procedure di versamenti e norme che attuano sentenze della Corte costituzionale con riferimento ad una intercettazione surrettizia di parlamentari o aventi carattere casuale. Ci sono variazioni in materia di protezione di dati personali e ipotesi disciplinari per i magistrati in caso di inserimento in un provvedimento di circostanze relative a fatti personali di terzi estranei, irrilevanti ai fini processuali; inoltre, la disciplina transitoria che prevede l'applicazione ai procedimenti in corso di alcune norme, il rinvio di un anno dell'entrata in funzione del tribunale del capoluogo di distretto l'applicazione della vecchia normativa per le procedure con autorizzazioni già emesse, ma che non possono durare comunque oltre 75 giorni, e l'entrata in vigore delle norme sui centri di intercettazione dopo tre mesi dall'entrata in vigore della legge.

è da diversi anni che il dibattito politico e parlamentare sottolinea l'esigenza di una modifica della disciplina delle intercettazioni telefoniche essendo venute più volte in evidenza alcune criticità nel loro utilizzo e nella loro diffusione. L'interesse di gran lunga prevalente, che ha mosso gran parte delle forze politiche di entrambi gli schieramenti, è stato quello della tutela della riservatezza delle persone,

di tutelare l'immagine, l'onorabilità e la *privacy* di chi, legittimamente, abusivamente o casualmente captato nei colloqui telefonici, si fosse ritrovato esposto alla dannosa pubblicità della propria vita privata sui mezzi di comunicazione a grande diffusione. Occorreva, quindi, un intervento legislativo non semplice, perché il diritto costituzionalmente garantito alla tutela della vita privata e alla libertà e segretezza delle comunicazioni essere bilanciato con altri precetti, di uguale rango costituzionale, quali quelli della libertà di stampa e del diritto di/alla informazione, dei principi dell'obbligatorietà dell'azione penale, del giusto processo e del dovere dello Stato di garantire ai cittadini la sicurezza personale. L'auspicato intervento riformatore si è rivelato vieppiù complesso in virtù della necessità di non derogare, attenuare o compromettere alcuni dei suindicati principi a discapito di altri, non soltanto perché la lesione di uno di essi si porrebbe ovviamente in contrasto con la Carta costituzionale, ma anche perché solo il loro integrale rispetto da attuare con un assetto normativo armonico costituisce garanzia di rispetto dei principi di democrazia, di libertà, di legalità e dei diritti dei cittadini alla corretta e integrale informazione alla sicurezza e al rispetto dei loro diritti soggettivi, individuali e collettivi. L'intervento normativo si è rivelato ancor più difficile in presenza delle note anomalie del sistema d'informazione nel nostro Paese, del rilevante tasso di criminalità organizzata e di reati contro la pubblica amministrazione e della difficoltà, in atto da molti anni, nei rapporti tra la magistratura inquirente e i titolari di funzioni pubbliche, elettive e non. Ci provò il Governo Prodi nella passata legislatura con un suo disegno di legge, che fu approvato, lo ricordo ai colleghi, dalla Camera dei deputati quasi all'unanimità, con sole sette astensioni, peraltro in gran parte della maggioranza dell'epoca, e con la convergenza dei Gruppi dell'attuale maggioranza di centrodestra, del nostro Gruppo, di quello dell'Italia dei Valori e di altri, che realizzava in tal modo un'accettabile equilibrio tra i valori e gli interessi in gioco. Ci hanno provato diversi Gruppi e singoli parlamentari in questa legislatura con diversi disegni di legge aventi un contenuto tra loro divergente, fino a quando l'attuale Governo ha deciso di presentare un suo disegno di legge, quello di cui stiamo discutendo, già esaminato

Casson, Finocchiaro e altri, e l'Atto Senato n. 781, a firma Della Monica e altri, di contenuto sostanzialmente analogo. Le proposte del nostro Gruppo avevano esattamente l'ambizione di affrontare e risolvere i problemi che ho evidenziato all'inizio, relativi alla tutela della riservatezza delle persone, all'eliminazione degli abusi nell'uso e nella diffusione delle intercettazioni, salvaguardando appieno la libertà di stampa e il diritto all'informazione, al pieno e corretto utilizzo di tale importante strumento di ricerca della prova nell'azione di contrasto alla criminalità comune e organizzata, a responsabilizzare in capo ad un magistrato inquirente e al personale a ciò delegato nell'obbligo di non diffondere le intercettazioni prima che esse diventassero pubbliche sulla base delle regole processuali, della distruzione e del divieto di diffusione delle comunicazioni irrilevanti per le indagini. Una linea di intervento, la nostra, chiara,

inaccettabile e peggiorativo financo del testo licenziato in prima lettura dalla Camera. Riassumo i punti, che ci sono ormai noti, per noi inaccettabili, per modificare i quali ci batteremo con determinazione con i nostri emendamenti e con la forza dei nostri argomenti, che trovano un ampio consenso nel Paese, nonché ricorrendo a tutti gli strumenti regolamentari a nostra disposizione. Innanzitutto vengono posti limiti e condizioni di ammissibilità delle intercettazioni del tutto inaccettabili. L'articolo 1, comma 10, rappresenta un superamento solo apparente, ma non reale, del richiamo agli «evidenti indizi di colpevolezza» quale presupposto per l'autorizzazione delle intercettazioni. Di fatto, si reintroduce tale improprio requisito di legittimità in forma di presupposti individualizzanti e di parametro interpretativo alla cui stregua il giudice deve valutare la sussistenza di «gravi indizi di reato». L'attribuzione al giudice collegiale del tribunale distrettuale della competenza ad autorizzare le intercettazioni determinerà non solo la paralisi degli uffici giudiziari distrettuali, ma paradossalmente favorirà le fughe di notizie in violazione della *privacy*, in quanto gli atti di indagine saranno messi a disposizione di un numero più esteso di persone e dovranno viaggiare non poco per raggiungere la destinazione. Inoltre, l'attribuzione al giudice collegiale della competenza ad autorizzare le intercettazioni è chiaramente asistematica, considerando che il giudice monocratico oggi, a legislazione vigente, non solo può disporre misure cautelari personali, ma anche irrogare un ergastolo, in sede di rito abbreviato. Ancora, la previsione dell'assenso scritto del procuratore della Repubblica, quale condizione di ammissibilità della richiesta di intercettazione da parte del pubblico ministero, con inevitabili ricadute negative sulle indagini e sull'efficienza dell'amministrazione della giustizia, costituisce un evidente ulteriore passo verso la gerarchizzazione delle procure. Altresì gravemente lesiva dell'azione investigativa è la prevista limitazione temporale della durata delle operazioni captative, eccessivamente restrittiva e del tutto inadeguata alla complessità di accertamento di taluni reati. Altrettanto irragionevole appare il divieto di utilizzazione delle intercettazioni in altri procedimenti o anche nello stesso procedimento, qualora il fatto sia diversamente qualificato e per esso non ricorrano i presupposti per per disporre le intercettazioni. Si consideri, inoltre, che la esclusione dei soli reati distrettuali dalla disciplina dei limiti di durata e dei presupposti delle intercettazioni è del tutto insufficiente, in quanto le intercettazioni per i reati cosiddetti satellite sarebbero comunque con le conseguenze immaginabili. L'estensione a tutte le intercettazioni ambientali, a prescindere dal luogo in cui si svolgano, del requisito della necessaria finalizzazione alla osservazione dell'attività criminosa in corso, oltre a depotenziare le attività di indagine, comporterà che non sarà mai possibile ottenere autorizzazioni ad intercettazioni ambientali per indagare su un reato già commesso, sia esso anche un omicidio o una strage. Un'assurdità palese anche per un'altra ragione: l'autorità giudiziaria, come ci è noto, indaga per definizione sui reati già commessi, quasi mai per finalità di prevenzione. Un chiaro *vulnus* al principio di ragionevolezza deriva dall'equiparazione alle intercettazioni, quanto al regime di ammissibilità, dell'acquisizione dei dati di traffico telefonico o telematico, che in quanto relativa ai soli dati "esterni" e non invece al contenuto delle comunicazioni, non può in alcun modo essere assistita dalle stesse garanzie, questo tipo di attività di indagine, né essere soggetta alle medesime limitazioni previste per le intercettazioni. La disposizione volta a sanzionare con la reclusione da 6 mesi a 4 anni l'utilizzo di registrazioni (effettuate fraudolentemente) di conversazioni alle quali l'autore abbia partecipato o sia stato presente (emendamento cosiddetto D'Addario), priva i cittadini della stessa possibilità della tutela giurisdizionale dei diritti, in violazione anche dell'articolo 24 della Costituzione, in quanto consente di utilizzare le suddette registrazioni solo "nell'ambito" di procedimenti giurisdizionali e non anche nelle fasi precedenti, quando cioè si debbano acquisire prove per denunciare, ad esempio, un estorsore o uno *stalker*. Nel contesto delle innovazioni che ho ricordato, particolare preoccupazione destano la procedura di ammissione, i limiti temporali di durata e la quasi soppressione di fatto delle intercettazioni ambientali. L'attribuzione al tribunale del capoluogo di distretto del potere autorizzatorio, seppur differito di un anno, implicherà un accrescimento di incombenze burocratiche e di passaggi procedimentali di enormi proporzioni. L'autorizzazione all'utilizzo dello strumento di indagine delle intercettazioni dovrà essere scritta e motivata dal pubblico ministero, dovrà essere condivisa e sottoscritta dal capo dell'ufficio, inviata unitamente all'intero fascicolo delle indagini al tribunale competente, a volte distante centinaia di chilometri, con dispendio di risorse e di tempo Un numero incalcolabile di magistrati inquirenti e giudicanti, di personale delle cancellerie e coadiuvanti, di autisti maneggerà le richieste e i fascicoli, li trasporterà, li depositerà occupando un tempo di lavoro enorme e rendendo oggettivamente concreto il rischio della violazione del segreto, con la paradossale conseguenza che la tutela della riservatezza sarà più a rischio in futuro rispetto alla Gruppi PD e IdV).* Altro che tutela della *privacy*! Il tutto per attuare un principio di controllo *ex ante* delle condizioni di ammissibilità che sarebbe molto più semplicemente conseguibile con altre più ragionevoli misure che abbiamo puntualmente proposto. Relativamente alla previsione della ristretta durata delle attività di indagine per rimediare ad un'estensione a volte irragionevole e costosa delle operazioni captative, si introducono limitazioni temporali inaccettabilmente brevi che di certo non coincideranno con la tempistica imprevedibile nella commissione dei reati, rendendo così le indagini casuali o inefficaci. Che cosa accadrà se le attività criminose si consumeranno dopo l'ora x di scadenza della possibilità di intercettare è facile immaginarlo. Così come è facile prevedere che con i sofisticati sistemi a disposizione della criminalità, i tempi di commissione dei delitti saranno parametrati ai rischi di essere intercettati o meno entro i limiti temporali prefissati autolesionisticamente dal legislatore. E non si dica, come ha fatto poco fa il relatore, senatore Centaro, che tali rischi non valgono per i reati di mafia e terrorismo. Costituisce un dato notorio volte durante le indagini si perviene all'individuazione delle attività illecite proprie della criminalità organizzata attraverso l'accertamento di reati comuni, quali le estorsioni, l'usura, le truffe, il traffico di stupefacenti e molti altri reati. Comprimere in misura così vistosa le indagini su tali reati significa fare un regalo alle bande criminali organizzate. Risibile, se non fosse che si tratta di questione molto seria, è la soluzione adottata per limitare le intercettazioni ambientali, uno strumento di indagine molte volte prezioso e risolutivo per l'accertamento di gravi reati. Subordinare il ricorso a tale strumento alla condizione che nel luogo si sta commettendo un reato significa annullare di fatto la possibilità di disporre intercettazioni ambientali. Particolarmente gravi sono le disposizioni che riguardano la libertà di stampa e il diritto dei cittadini all'informazione. Sul punto cruciale relativo alla libertà di informazione, la prima significativa limitazione del diritto di cronaca deriva dall'inasprimento irragionevole delle pene per la rivelazione illecita di atti coperti da segreto o per la pubblicazione arbitraria di atti processuali, nonché dall'estensione della responsabilità da reati agli enti (in particolare gli editori dei giornali), che possono giungere - o potevano, secondo il testo della Commissione - fino a 464.000 euro, limite massimo che la maggioranza oggi propone di ridurre con apposito emendamento dopo le note proteste degli editori. Ma la modifica più significativa nel testo licenziato dalla Commissione riguarda la disposizione di cui all'articolo 1, comma 5, che precludeva finanche la pubblicazione per riassunto degli atti di indagine, ancorché non più coperti da segreto, fino alla conclusione delle indagini o al termine dell'udienza preliminare. Tale *vulnus* del diritto all'informazione era peraltro aggravato dal divieto, di cui all'articolo 1, capoverso 2-*ter*, della pubblicazione, anche per riassunto o nel contenuto, delle richieste e ordinanze emesse in materia di misure cautelari, della documentazione e degli atti relativi ad operazioni captative anche laddove non sussista il segreto investigativo, così precludendo totalmente la cronaca giudiziaria relativamente a fatti di interesse pubblico evidente. A fronte della gravità e abnormità di tali disposizioni e dopo la generalizzata protesta della stampa italiana, la maggioranza si è orientata (correndo ai ripari, dal suo punto di vista) a tornare, con una delle proposte emendative presentate, al testo della Camera consentendola pubblicazione per riassunto, il che attenua ma non elimina affatto la grave lesione alla libertà di stampa. I suddetti divieti appaiono tanto più incompatibili con gli articoli 21 europea dei diritti umani ove si consideri il rilevante inasprimento sanzionatorio previsto dal testo per i reati in materia di pubblicazione degli atti, che rischia di inibire del tutto la libertà di stampa e, quindi, di privare i cittadini del diritto a ricevere informazioni su fatti

giustificarsi neppure in ragione dell'esigenza di tutelare beni giuridici di rilievo costituzionale e che appaia nettamente contrasto appunto con gli articoli 21 della Costituzione e 10 della Convenzione europea dei diritti umani e funzionale soltanto a privare i cittadini del diritto all'informazione. Altre disposizioni molto discutibili sono quelle relative alle intercettazioni indirette e casuali a carico dei parlamentari e loro collaboratori, alla speciale disciplina prevista per gli agenti dei servizi, all'introduzione dell'astensione obbligatoria del giudice e sostituzione del PM che abbiano pubblicamente rilasciato dichiarazioni concernenti il procedimento affidatogli, alla fissazione di tetti di spesa per le intercettazioni ripartiti tra il livello nazionale, distrettuale e circondariale e altre disposizioni minori. Questi tetti di spesa determineranno il fatto che settembre, a ottobre o a novembre non si potranno fare più intercettazioni. Alle gravi preoccupazioni espresse da noi e provenienti dal Paese, la maggioranza e il Governo hanno tentato di porre rimedio con gli emendamenti depositati nei giorni scorsi in vista dell'avvio della discussione in Aula. Senonché, alle limitate e insufficienti proposte in senso migliorativo del testo licenziato dalla Commissione, quasi del tutto coincidenti con il ripristino del testo approvato in prima quella relativa alla riscrittura delle disposizioni transitorie, che rischia se approvata di far saltare o, nella migliore delle ipotesi, aggravare un numero non quantificabile di procedimenti pendenti. È facile immaginare la carica demolitrice di tale abnorme disposizione, contrastante, come mai avvenuto prima, con il principio del *tempus regit actum* in un numero enorme di procedimenti, compresi quelli di più stringente attualità relativi a diffusi fenomeni di corruzione, che tanto sconcerto hanno determinato nell'opinione pubblica. E quali effetti produrranno le norme restrittive del diritto di cronaca sugli atti già resi pubblici o disponibili ai difensori delle parti? Dunque, il testo e gli emendamenti che la maggioranza e il Governo chiedono a quest'Aula di approvare in questi giorni costituiscono un pasticcio normativo, con disposizioni confuse e dannose, che castrano irrimediabilmente efficaci strumenti di indagine, che affievoliscono in modo inaccettabile il diritto all'informazione, come mai era avvenuto nella nostra storia repubblicana, e che oggettivamente renderanno più agevole delinquere e più difficile scoprire e perseguire e perseguire chi delinque. La realtà, signor Presidente, è che di fronte a noi vi erano, e vi sono, due linee chiare per affrontare e risolvere problemi che esistono: esistono: quella di limitare fortemente le intercettazioni e, quindi, l'efficacia delle attività di indagine, con oggettivo indebolimento della sicurezza dei cittadini e del contrasto alla criminalità di ogni genere, di stampa, o, in alternativa, quella di vietare e bloccare la diffusione delle intercettazioni abusive o estranee alle indagini e ai procedimenti penali, responsabilizzando e sanzionando magistrati, polizia giudiziaria e personale per la violazione del segreto d'ufficio e la strumentalizzazione nell'uso e nella diffusione delle intercettazioni non rilevanti per fini di giustizia, in tal modo tutelando la riservatezza dei cittadini e la corretta ed efficiente amministrazione della giustizia. con forza questa seconda linea, che rappresenta ciò che i cittadini chiedono. Voi avete scelto la prima strada, quella che indebolirà ulteriormente il nostro già collassato sistema giudiziario e costituirà il più grave attacco alla libertà di stampa mai concepito nella storia Ecco perché abbiamo il dovere sacrosanto di contrastare in ogni modo questo disegno di legge, con tutti i mezzi democratici a nostra disposizione in Parlamento e nel Paese.

Non ci avete voluto ascoltare, non avete inteso accogliere neanche le più ragionevoli delle nostre proposte. Avete scelto di tirare dritto, di sconquassare l'impianto investigativo del nostro Paese, che si è consolidato e perfezionato nel corso degli anni e di cui pure il Governo si vanta in coincidenza di questa o quella operazione di cattura di latitanti o di operazioni di polizia particolarmente incidenti attività criminose. Non ci avete voluto ascoltare, e non avete ovviamente voluto ascoltare l'allarme di tutta la magistratura. Ascoltate almeno il serio e fondato allarme del Procuratore nazionale antimafia, di tutte le forze di polizia, di tutti i giornalisti, degli editori, degli scrittori, degli intellettuali del nostro Paese e, soprattutto, delle vittime dei reati. Se non lo farete, vi assumerete una gravissima responsabilità nei confronti dell'intero nostro Paese. *(Applausi

la materia della quale ci stiamo occupando, dal momento che nel corso di questi ultimi anni le cifre, ballerine, hanno evidenziato realtà esattamente contrarie ai dati ufficiali. Il numero dei decreti intercettativi nel nostro Paese, in base ai dati conosciuti recenti, è di 130.000. Il decreto Il decreto è collegato a ogni singola utenza e deve essere rinnovato, a legislazione vigente, ogni 15 giorni. Sicché il numero delle persone intercettate è stimato

così come evidenziato dalle sentenze nn. 416 e 450 del 2000 della Corte costituzionale. Prima questione: violazione degli articoli 21 e 117 della Costituzione (in riferimento al rispetto degli obblighi internazionali,

Ovviamente noi terremo conto in questa nostra discussione anche degli emendamenti presentati dalla maggioranza. Qualora fosse approvato l'emendamento della maggioranza contenente il ripristino della «possibilità di pubblicazione per riassunto degli atti non più coperti da segreto», non avrebbe alcun fondamento la previsione del divieto di pubblicazione in qualsiasi forma (parziale, per riassunto o nel contenuto) degli atti relativi a conversazioni o a flussi del traffico telefonico. Invero, se l'atto non è più coperto dal segreto e se gli atti non coperti dal segreto sono sempre pubblicabili per riassunto, il divieto solo per una categoria di atti si configura quale censura per la stampa. Il comma 2 dell'articolo 21 della Costituzione afferma il principio per il quale «La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure». Incide, inoltre, sull'articolo 21 della Costituzione il divieto di ripresa audiovisiva dei dibattimenti, qualora una parte non consenta non solo alla ripresa della propria immagine, ma alla ripresa audiovisiva del processo e anche alla trasmissione radiofonica, alla ripresa delle immagini fotografiche e alla registrazione fonografica. Sembra di compiere un salto indietro di ottant'anni: sembra di essere tornati al diritto di cronaca di regime. Ancora oggi noi parliamo di Gino Girolimoni, distrutto da un'inchiesta di regime e condannato a vita come pedofilo assassino, mentre era innocente, perché la stampa, per non disturbare il regime, non diede notizia della sua assoluzione! Ancora oggi nel nostro Paese si parla di Girolimoni! Ricordiamoci a cosa serve la stampa in un regime di democrazia e di libertà! Seconda questione: è irragionevole la previsione di durata massima delle intercettazioni telefoniche, sia che si tratti di omicidio, di una strage, di un'ingiuria, di delitti di criminalità organizzata o di traffico di rifiuti pericolosi, di un reato punito con l'ergastolo o di un reato punito con la multa sino a 516 euro. reati per i quali sono previsti tempi differenziati di durata delle indagini, da sei mesi a due anni: per tutti si prevede però lo stesso termine di durata delle intercettazioni, per l'ingiuria e per la strage.

vi è la possibilità di una proroga di 15 giorni quando «emerge l'esigenza di impedire che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero che siano commessi altri reati». Invero, siffatta previsione di proroga limitata a 15 giorni contrasta, qualora permangano le condizioni della proroga, ossia la necessità di impedire che un'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori (pensiamo ad un sequestro di persona con il sequestrato nelle mani dei sequestratori), con l'articolo 3 e l'articolo 117 della Costituzione, che assegna allo Stato il compito di garantire con adeguata e coerente legislazione i diritti dei cittadini, l'ordine pubblico e la sicurezza. Si pensi alla vittima del reato, si pensi al sequestrato nelle mani dei sequestratori che confida nello Stato e nei suoi organi e che invece dovrà subire la vergognosa previsione secondo cui,

la durata delle intercettazioni è pari alla durata delle indagini. Se c'è un sequestro di persona senza richiesta di riscatto, ovvero si sconosce la ragione del sequestro, la durata delle intercettazioni non potrà superare i 75 giorni. È come stabilire per legge che, verificatasi una calamità naturale, lo Stato ricercherà le vittime sotto le macerie solo per tre giorni, perché oltre tale tempo è statisticamente improbabile che la vittima sia ancora viva.

«Negli stessi casi di cui al comma 1 è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti solo se vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa». se viene trovato il cadavere di una persona assassinata le ambientali potranno farsi solo se in un luogo individuato «si stia svolgendo l'attività criminosa». È un paradosso: invero, l'omicidio è già avvenuto, ma l'indagine sull'omicidio può farsi ricorrendo alle ambientali solo se vi è fondato motivo di ritenere che si stia svolgendo un altro reato. Anzi, secondo la lettura della norma, se sia in corso l'attività criminosa per la quale si indaga, ossia un omicidio (con un cadavere crivellato di colpi) di colpi) che si protrae nel tempo. Ma tutto ciò, comunque, per 75 giorni. In tal modo l'intercettazione ambientale viene svuotata del suo fine strumentale (mezzo di ricerca della prova), divenendo una cosa diversa, collocabile parzialmente nello schema dell'articolo 55 del codice di procedura penale («la polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercare gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quanto altro possa servire per l'applicazione della legge penale»). Il «deve», previsto dall'articolo 55 del codice di procedura penale, rispetta il principio costituzionale previsto dall'articolo 112 della Costituzione (azione penale obbligatoria) che, invece, viene così violato, come è violato l'articolo 117 della Costituzione (lo Stato deve legiferare per assicurare l'ordine pubblico e la sicurezza). Quinta questione: è incostituzionale, per violazione dell'articolo 111 della Costituzione («la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa») la proposta di modifica dell'articolo 292 del codice di procedura penale (ordinanza di cattura). comma 18, del disegno di legge: «Nell'ordinanza le intercettazioni di conversazioni, comunicazioni telefoniche o telematiche possono essere richiamate soltanto nel contenuto e sono inserite in un apposito fascicolo allegato agli atti». Il successivo comma 19 precisa che «In ogni caso i difensori possono prendere visione del contenuto integrale dell'intercettazione, richiamata nell'ordinanza per l'applicazione delle misure». la facoltà di consultazione da parte del difensore implicitamente presuppone l'incompletezza e la genericità dell'ordinanza che dispone l'arresto,

Invero non potrà esservi una motivazione, non potendo il giudice esprimere le sue valutazioni in ordine ad una o più intercettazioni poste a carico dell'arrestato, potendo solo richiamarle genericamente nell'ordinanza. La parola «contenuto» significa «riferimento generico privo di riscontri documentali» (così la relazione al progetto del codice di procedura penale). Per la giurisprudenza la valutazione è «verifica del contenuto di una prova, della rilevanza e della fondatezza». Sicché, una persona viene arrestata in forza di un provvedimento con motivazione generica ed inespressa. La facoltà concessa al difensore di «prendere visione integralmente della intercettazione richiamata nell'ordinanza» non garantisce l'imputato arrestato 104 del codice di procedura penale, abbia imposto il divieto di conferire dell'avvocato con il suo assistito. L'interrogatorio dell'arrestato deve essere compiuto entro cinque giorni (riducibili a due); sicché, l'imputato verrà sottoposto all'interrogatorio senza conoscere nello specifico le prove a suo carico e le valutazioni del giudice. Ciò contrasta con l'articolo 111 della Costituzione e con il diritto di difesa, anche in considerazione del fatto che l'interrogatorio di garanzia è finalizzato a verificare le condizioni

si applicano le disposizioni di cui agli articoli 192, commi 3 e 4, 195 comma 7, e 203». I commi 3 e 4 dell'articolo 192, riguardano la valutazione delle «dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato» o dell'imputato in procedimento connesso La griglia di valutazione dei «gravi indizi di reato», indicata nel disegno di legge riporta così ai criteri di valutazione dei gravi indizi di colpevolezza. Semmai la griglia da richiamare era quella del comma 2 dell'articolo 192, ossia: «L'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi non siano gravi, precisi e concordanti».

Ora, con l'abrogazione che è stata proposta, si sposta esclusivamente alla tutela per i reati di mafia, ma vengono esclusi i reati di criminalità organizzata, le varie bande che operano nel nostro Paese, che rientrerebbero così nella procedura normale ossia nei limiti e nei presupposti intercettativi. Si tratta di un'irragionevole abrogazione di un articolo fondamentale voluto da Giovanni Falcone per la lotta al crimine organizzato: tutto il crimine organizzato. È poi assolutamente irragionevole la norma transitoria che prevede nell'ambito dello stesso procedimento che ci siano intercettazioni eseguite con l'applicazione della normativa vigente, intercettazioni che hanno i presupposti della normativa vigente ma i tempi della normativa introducenda e intercettazioni che hanno sia i presupposti che i tempi nuova normativa. In questo modo, altro che principio del *tempus regit actum*! Questo è il caos della normativa transitoria. Per questi motivi, chiediamo che non si dia corso, per manifesta incostituzionalità, all'esame del disegno di legge

Ho avuto un abbassamento di voce, ma non un abbassamento della mia volontà di esprimere un parere che esce un po' dal tema regolamentare, perché affronta una questione che credo stia in cima a tutti i nostri discorsi, a quelli odierni e a quelli che faremo. La pregherei di concedere che un paio di decibel in più mi aiutino a farmi capire meglio. sul «Corriere della Sera» un suo articolo che, prendendo le mosse dalla tragica vicenda di Walter Tobagi, affermava come egli avesse esercitato l'opera sua sul piano - forse addirittura più insidioso del diritto e dell'ordine pubblico - della cultura e dell'informazione, attraverso le armi dell'inchiesta e dell'analisi critica. Grazie di queste parole, che le fanno onore! onore! Signor Presidente, vorrei che questo suo condivisibile giudizio fosse d'introito ai lavori che concluderanno una grande e spero non inutile fatica, e che allo spirito delle sue parole l'Aula impronti le nostre prossime sedute. Rinnovo l'invito, per quel che posso, a far sì che prevalga quella ragionevolezza così spesso elusa, perché la ragione politica pretende che si privilegi un altro ragionamento. Basti pensare ai tagli inferti proprio alla cultura, cui si sta tentando di opporre *in extremis* qualche incerto e pericolante rimedio. So bene, signor Presidente, che non ci misuriamo con una di quelle congiunture in cui la storia assegna a tale questione un significato drammatico, ma il solo fatto di doverci riferire a un articolo della nostra Carta (parlo ovviamente dell'articolo 21) giustifica il malessere che ha accompagnato sin qui la disputa sulle intercettazioni. Quindi domando, signor Presidente, senza alcun intento polemico, perché, di fronte a un disagio di tale rilevanza (Benedetto Croce la chiamerebbe sofferenza etica), non abbiamo avvertito tutti insieme, maggioranza e minoranza, che questa sorta di spaesamento è in realtà al centro di una grande e grave questione democratica. Eppure siamo in un'Aula dove la libertà di stampa, anche quella che rischiasse la meno inquietante delle lesioni, dovrebbe avere il suo presidio più efficace e vincolante. Qui, per la natura del nostro stesso compito dovremmo essere indotti, nel nome di un bene che ci fa uguali, a volgere i nostri lavori in direzione di salvaguardie che superino, nell'interesse comune, le chiusure pregiudiziali e gli opportunismi politici, strutturali o contingenti che siano. Ciò, perché la libertà di espressione deve tendere alla promozione del confronto pubblico e della responsabilità personale, a tutelare i diritti di ciascuno e di tutti, a contrastare le invadenze dei poteri, a difendere la democrazia dalle intolleranze occulte e dalle aggressioni fin troppo evidenti e perché soltanto un giornalismo disposto a svolgere questo compito è lo strumento garante della politica, mentre in caso contrario può essere solo il suo servo. C'è chi risolverebbe alla svelta il problema: gli basterebbe ridurre la politica al minimo, opponendole diffidenza e disinteresse e magari rivolgendo qualche anacronistica minaccia normativa a un giornalismo che interpreti - mai che ometta - i suoi doveri deontologici. Non posso dimenticare, signor Presidente, Albert Schweitzer che, nel suo celebre lebbrosario di Lambaréné, mi disse: «Fino a quando non diremo cose che a qualcuno dispiaceranno non diremo mai per intero la verità». Del resto, ricorderete come Orwell immaginasse un Ministero della verità il quale avrebbe provveduto a cancellare quotidianamente i fatti scomodi, distruggendo i segni che essi lasciano. La cupa profezia si è posta da allora come un'epigrafe in testa al nostro modo di intendere l'informazione, la sua natura e il suo scopo in una società liberale e riformista, per ricordarci che la democrazia va difesa ogni giorno. Forse, per comprendere che cosa è realmente in gioco vale la pena di ricordare anche quanto ha detto Hans Magnus Enzensberger: «Ai giornalisti di oggi spetta non il dovere, ma certamente il compito di fare chiarezza su tutto quanto, per loro merito o demerito, ci coinvolge»; aggiungervi il giudizio di Amartya Sen, premio Nobel per l'economia, che ha avuto l'ardire, oltre che l'umiltà, di considerare l'informazione oggi più importante persino dell'economia: un azzardo - direte - ma non privo di qualche fondamento. Giorni fa in un giornale ho scritto a proposito del cartello appeso al collo di un partecipante al *sit in* davanti a Montecitorio in cui si leggeva "Io non ho paura, intercettatemi": come a dire che questo disegno di legge favorisce chi ha colpe o reati da nascondere. Era una posizione di rifiuto totale, estrema, e quindi a sua volta contestabile. Basta infatti approfondire il problema, in cui si affrontano due diritti fondamentali (l'informazione dovuta da una stampa libera e quella che viola gratuitamente la riservatezza personale) per rendersi conto della profonda differenza, in questa delicata materia, tra chi è investito di responsabilità pubbliche, sia elettive che conferite dallo Stato, e un semplice cittadino. anziché tentare una equilibrata composizione, difficile ma necessaria, si è scelta la strada, a prima vista più facile, di restringere al massimo le intercettazioni, ricorrere alla minaccia del carcere per i giornalisti (poi ragionevolmente lasciata cadere), infliggendo multe pesantissime, anche se poi ridotte per le piccole testate, a carico degli editori, aprendo la strada all'intervento della proprietà sul contenuto dei giornali è competenza esclusiva del direttore. Una serie di errori non da poco, ancora passibili di correzione, conferisce qua e là un carattere repressivo e illiberale a questo progetto, e lo sarebbe ancora di più se la pratica delle intercettazioni dovesse limitare l'azione legittima e indispensabile della magistratura, per esempio - cito il caso più vicino e irrisolto quando la comunità nazionale si sente offesa dalla cosiddetta cricca (una parola d'uso comune per indicare un clima ben più che equivoco). Qui la materia affronta aspetti controversi di legittimità che affido a chi ha dottrina per farlo; ma sono persuaso signor Presidente, che in un Paese in cui dopo 21 anni si vanno a cercare le impronte lasciate dagli attentatori di Giovanni Falcone sugli scogli dell'Addaura e dove, rovistando tra vecchie collezione di giornali, si trova la fotografia di un agente segreto sempre presente quando è alle viste o in preparazione o addirittura in atto un'azione eversiva gravemente criminosa, la funzione della stampa si riveli fondamentale. Perciò, lungi dal restringerne le facoltà, va ricercata e perseguita la sequela di reticenze, ambiguità e fellonie, se non si vuole coprire una manifesta e impunita lesione della nostra stessa legittimità democratica. Mi limito a citare le parole di un nostro collega della passata legislatura, l'autorevole ed equanime Andrea Manzella: il messaggio complessivo è che la lotta al crimine in Italia, terra di molte mafie e di molte complicità, sarà indebolita. Ribassi di pene per non reati, cioè per la libertà giornalistica di informare su atti non più segreti, non servono a cancellare il nonsenso strutturale dell'intero progetto,

il luogo della nostra risposta a una delega popolare fondata sul valore e sulle modalità della trasparenza politica, civile e morale, non può non disporsi a compiere un dovere di inestimabile significato. E perché nessuno si senta escluso dalla vitale necessità di salvaguardare il dettato costituzionale, lasciatemi ricordare la parola più alta, data a tutti perché venga pronunciata per tutti. Una parola che vive dentro e fuori di noi, quand'anche non ci si accorga della sua presenza. Una parola che è come l'aria, la quale ci tiene in vita, si può dire, quasi a nostra insaputa, chiunque si sia e dovunque si stia. È una parola che va detta e udita in nome delle responsabilità che essa esige. Quella parola è così solenne che si stenta a ripeterla senza qualche imbarazzo, ma libertà - cui tutti dobbiamo continuamente richiamarci - è la prima a dar vita alle nostre speranze di non venire sconfitti dalle nostre stesse sordità, o peggio dalla nostra rassegnazione. Pronunciamola, dunque, dandole un fondamento comune: è la sola che nessuno può pronunciare solo per se stesso, ed è di quelle che, signor Presidente, in quest'Aula devono avere la precedenza. *(Vivi,

abbiamo tutte le migliori intenzioni di continuare la nostra battaglia parlamentare, con gli strumenti parlamentari di cui disponiamo. In questa fase, teniamo a sottolineare che sono almeno nove i profili di illegittimità costituzionale da cui è toccato il disegno di legge sono diversificati e riguardano aspetti relativi alla libertà di stampa, alla sicurezza dei cittadini e alla tutela della riservatezza dei cittadini. Mi limiterò ad accennare i profili di illegittimità costituzionale, poiché su questi punti interverranno i colleghi in maniera più dettagliata. Ricordo innanzitutto che il divieto di pubblicazione degli atti di indagine, ancorché non più coperti dal segreto, fino alla conclusione dell'indagine o al termine dell'udienza preliminare si presenta come assolutamente incompatibile con il diritto di informazione e con il diritto all'informazione di cui all'articolo 21 della Costituzione, all'articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e all'articolo 10 della Carta di Nizza. Situazione che, per quanto riguarda la libertà di pubblicare, è vieppiù aggravata dal divieto di pubblicare tutta una serie di atti di interesse collettivo, soprattutto per quanto concerne fatti di rilevante interesse pubblico. Il *blackout* informativo che entrerebbe in vigore con questo disegno di legge contrasta, oltre che con le norme della Costituzione e con quelle di diritto europeo e internazionale che ho ricordato, con le sentenze della Corte di Strasburgo dei diritti dell'uomo. Quest'ultima è intervenuta ripetutamente in anni recenti per affermare come fondamentale il diritto dei giornalisti a fornire e del pubblico a ricevere notizie di cronaca giudiziaria. Questo diritto dei giornalisti e, di converso, dei cittadini è ritenuto prevalente finanche sulla *privacy* degli interessati e sul segreto istruttorio. La Corte di Strasburgo è intervenuta in diverse occasioni. Ricordo solo il caso Dupuis e Pontaut, in cui è stata condannata la Francia, la quale, a sua volta, con la sua magistratura, aveva condannato alcuni giornalisti che si erano limitati a citare fatti e notizie relativi a servizi segreti francesi e ad indagini che lambivano il Presidente della Repubblica francese. Ora, la Corte europea di Strasburgo ci ricorda come la stampa possa essere definita per così dire il *chien de garde*, ossia il cane da guardia della democrazia e - aggiungo io - del corretto svolgimento delle attività della magistratura. Ci sono però altri aspetti che presentano profili di illegittimità costituzionale. Uno di questi riguarda le sanzioni che vengono irrogate ai giornalisti: la sanzione del carcere, ancora ribadita, è assolutamente sproporzionata condannata dalla Corte europea di Strasburgo. Allo stesso modo le sanzioni sproporzionate a livello di ammenda sono ritenute assolutamente in contraddizione con l'articolo 10 della Convenzione europea, proprio perché tra il diritto del cittadino a sapere e del giornalista a scrivere e, dall'altra parte, il diritto dei cittadini a sapere tutto rispetto anche al segreto istruttorio deve prevalere il diritto della collettività. Altri punti che presentano problemi di illegittimità costituzionale concernono la sospensione obbligatoria - così come prevista dal disegno di legge Alfano - del giornalista e le norme che hanno a che fare con "l'emendamento D'Addario", le quali si accaniscono su particolari categorie di giornalisti, che sono quelli non professionisti, non iscritti all'albo dei giornalisti. Ricordiamo, invece, come il giornalismo di inchiesta sia caratterizzato soprattutto dalla presenza di giovani giornalisti, giornalisti *freelancer*, i quali sono spesso giornalisti pubblicisti non ancora iscritti all'albo. Questa discriminazione costituisce un chiaro sintomo di illegittimità costituzionale. Altro punto concerne il divieto di riprese fotografiche e televisive dei dibattimenti e delle relative trasmissioni, secondo modalità che contrastano con l'articolo 21 della Costituzione e l'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti umani. che, nel delineare uno dei cardini del giusto processo di cui all'articolo 111 della Costituzione, rappresenta un principio essenziale di ogni ordinamento democratico. Ci sono poi due interventi all'interno del disegno di legge che prospettano ulteriori profili di illegittimità costituzionale. Si tratta di un allargamento di prerogative di immunità, per così dire, riguardanti gli appartenenti ai servizi di informazione e sicurezza e concernenti le intercettazioni nei confronti di coloro che stanno attorno al parlamentare: così come sono scritte, le norme configurano dei privilegi assolutamente inaccettabili, anche per quanto riguarda l'allargamento della sfera di immunità dei parlamentari. Noi non condividiamo norme di tal genere, ma, quand'anche si volessero approvare, bisognerebbe farlo con legge di rango costituzionale. L'ultimo punto concerne la sicurezza dei cittadini e i poteri limitati relativi alle investigazioni della polizia e della magistratura. Il disegno di legge Alfano non solo introduce misure lesive della libertà di stampa, ma prevede anche una significativa limitazione dei poteri investigativi della magistratura, con particolare riferimento ai tabulati, alle videoriprese, ai requisiti di ammissibilità dell'istituto delle intercettazioni, all'imposizione di un collegio per intervenire quando si debba decidere per una intercettazione di questo tipo, all'inutilizzabilità

di recente dagli operatori del settore sicurezza e giustizia, da tutti i sindacati di polizia di qualsiasi estrazione e finanche dal procuratore nazionale antimafia e dal capo della polizia. Queste limitazioni, in particolare quella relativa ai termini massimi di durata delle operazioni captative, non solo privano di strumenti di indagine preziosi gli organi inquirenti, ostacolando l'attività di accertamento dei reati e così pregiudicando la tutela della sicurezza dei cittadini, ma non possono peraltro in alcun modo giustificarsi in nome della tutela della *privacy*. Allora, ancora una volta, dobbiamo affermare che questo disegno di legge, anziché tutelare la riservatezza dei cittadini, si configura prevalentemente ed essenzialmente come un disegno di legge che tende a bloccare le indagini della polizia e della magistratura, alla faccia della vostra decantata sicurezza dei cittadini, e che mira ad imbavagliare la stampa.

e che arriva, nella sua pratica attuazione, a un risultato diverso: quello di costruire un testo palesemente in contrasto con la Costituzione, che non serve né ai magistrati per svolgere indagini secondo priorità e obiettivi investigativi e con le risorse necessarie a conseguire dei risultati, né ai cittadini per farsi scudo rispetto all'abuso delle intercettazioni e a tutto ciò

che parte proprio dal testo licenziato dalla Commissione: testo che - ricordo - doveva trovare un'ampia condivisione, nelle parole del relatore

della società e dei Gruppi parlamentari di opposizione. Il contributo, invece, lo ha dato solo il Popolo della Libertà con 11 emendamenti, tutti ripiegati all'interno di una trattativa estenuante, che continua

prevede che le norme relative alla ricusazione del giudice, alla sostituzione del pubblico ministero in udienza, alla tutela delle conversazioni e delle comunicazioni dei difensori, alle riprese in udienza dibattimentale siano immediatamente applicabili ai procedimenti in corso. Tutto questo è qualcosa di più e di diverso da ciò che abbiamo esaminato in Commissione. Altro che principi, di cui parlava prima il Presidente del Senato! Qui si tratta di una norma che stravolge, paralizza, demolisce e distrugge attività di indagine, procedimenti in corso, processi che si stanno celebrando. E tutto questo, operando una disparità di trattamento anche tra soggetti che nello stesso procedimento si trovano nella medesima condizione: ad essere più o meno sfortunati perché, a seconda di come e di quando temporalmente sono coinvolti nel procedimento, avranno una corsia e un binario diversi. tutto ciò con la certezza del diritto e - cari colleghi della Lega - con la certezza della pena, poco comprendiamo. Tutto questo ha invece molto a che vedere con la Costituzione e con la violazione di una serie di norme che non guardano solo, come alcuni hanno detto in precedenza, alla tutela corporativa di una parte dell'ordinamento, quello giudiziario. Quando diciamo che il pubblico ministero può essere sostituito in udienza se risulta iscritto nel registro degli indagati per il reato di cui al 379-*bis* del codice penale, quindi con riferimento agli atti del procedimento a lui assegnato, sostanzialmente introduciamo una norma che che cancella un intero processo perché consente la sostituzione del pubblico ministero per un fatto, l'iscrizione nel registro degli indagati, che, come è noto, è un atto dovuto. Come sia conciliabile tutto questo, da un lato, con l'articolo 27 della Costituzione (anche sul diritto di difesa del pubblico ministero, che si vede tolta l'indagine cui ha lavorato, magari per diversi anni, solo perché qualcuno

che presiedono anche all'efficienza e all'efficacia dell'azione amministrativa, da cui non è estranea - o non dovrebbe essere estranea - l'amministrazione della giustizia, come voi stessi dite, perché bisogna renderla manageriale, efficiente e così via) non lo abbiamo capito. con il principio fondamentale - che non è a garanzia del magistrato, ma del cittadino - della inamovibilità del magistrato e del giudice naturale precostituito per legge, ancora oggi non lo abbiamo ben chiaro, perché attraverso la possibilità di rimuovere il pubblico ministero solo perché iscritto nel registro degli indagati si costruisce un sistema che, alla fine, porta al risultato di non dare garanzia e certezza ai cittadini dell'impianto costituzionale che a presidio dei cittadini (e non dei magistrati) è stato organizzato e costruito.

credo che in questo Paese esista il problema dell'attuazione dei principi contenuti nell'articolo 2 della Costituzione, primo tra tutti il diritto alla riservatezza e alla *privacy*, che fa parte della tutela della dignità della persona umana. Ma se noi introduciamo questo principio, dobbiamo avere il coraggio introdurlo a tutto tondo, perché l'attività invasiva ed intrusiva della *privacy* dei cittadini non è solo ed esclusivamente collegata al tema delle inchieste e delle indagini giudiziarie (queste ne rappresentano una parte, non tocca a me dire se modesta o prevalente),

chissà come, si tuteleranno la riservatezza e questa parte dei diritti fondamentali della persona umana. Voi state facendo un'operazione che è ancora peggiore, perché non persegue e non raggiunge neanche l'obiettivo che voi dite di esservi prefissi, cioè quello di evitare il cosiddetto tritacarne mediatico-giudiziario (ormai siamo abituati a parlare per slogan e per schemi), perché voi introducete, di fatto e di diritto, un doppio regime di pubblicità. Infatti, quando dite che gli atti non sono più segreti - e non lo sono perché entrano nella sfera di conoscenza dell'indagato e quindi anche dei difensori - sono atti

da altri. Come dicevo, introducete un doppio regime perché prevedete comunque una pubblicità rispetto alla platea di soggetti che hanno accesso a quelle informazioni che voi definite riservate e che stanno nella fascia che va dalla *discovery* - e quindi dal superamento della fase della copertura del segreto - alla fase del rinvio a giudizio, dell'udienza e del dibattimento. In questa fase c'è una serie di privilegiati, di soggetti qualificati

degli atti e, quindi, della violazione del diritto, costituzionalmente garantito, alla riservatezza e ad evitare l'uso strumentale di informazioni riservate. Il problema infatti è che la pubblicazione sulla stampa di determinati atti viene interdetta perché si parte dal presupposto che vi sia un uso strumentale di quelle informazioni che, fornite ad una platea più ampia, possa - ed è ciò che in alcuni casi è avvenuto - ledere la libertà e la dignità della persona. Ma quale uso

qualificati interdetti dall'utilizzo di queste informazioni, pone anche il problema di una disparità di trattamento e di una violazione ancor più ampia delle norme costituzionali in materia di libertà di informazione e di manifestazione del pensiero. Inoltre, signora Presidente, non voglio

oggi opera contro la mafia. Anzi, crea un problema enorme perché non consente di svolgere, in tempi che siano in sintonia con le esigenze

non consente alle parti offese, alle vittime del reato, di poter accedere facilmente a questo strumento che, ancor prima che essere uno strumento in mano all'accusa, è uno strumento in mano alla difesa. Da ultimo, l'idea di aver l'idea di aver introdotto solo ed esclusivamente per le intercettazioni il regime autorizzatorio del tribunale collegiale è irragionevole e viola gli articoli 3 e 97 della Costituzione. Vi Mi volete spiegare come è possibile che un giudice monocratico possa anche in sede di rito abbreviato condannare all'ergastolo e per disporre le intercettazioni rispetto a quel procedimento debba chiedere agli insegnanti di sostegno? Sotto il profilo giuridico state facendo diventare - e di fatto è questa la più grande bomba dal punto di vista costituzionale - l'intercettazione,

Non parlo poi della norma sulle intercettazioni indirette ed occasionali che coinvolgono i parlamentari perché credo si commenti da sola e rappresenti la ciliegina sulla torta di un provvedimento che è incostituzionale e rispetto al quale, forse, sarebbe opportuno, signora Presidente, che non si disponesse alcun rinvio in Commissione. se si devono rinviare solo gli "undici comandamenti" del Popolo della Libertà per consentirgli di trovare al suo interno la quadra, forse è meglio licenziare questa schifezza oggi o domani, e poi alla Camera vedremo come, insieme alla ragionevole durata del processo, anche questa schifezza morirà.

i colleghi della maggioranza grazie al testo e agli emendamenti siano riusciti in una sorta di miracolo: abbiano cioè introdotto a Costituzione invariata il bicameralismo imperfetto a favore della Camera. infatti tali e tanti gli strafalcioni nel testo e negli emendamenti a spingere il Presidente della Camera a dire di mandargli il testo per farglielo correggere e poi rimandarlo qui per la lettura conforme. Mi complimento, perché forse non avremo più bisogno di rivedere

eviterei di addentrarsi eccessivamente perché non mi sembra particolarmente ferrato nella materia, viste le posizioni tenute su altri temi. Prendiamo atto che è stato introdotto questo bicameralismo imperfetto, come segnalava poco fa ironicamente anche il presidente D'Alia. il presidente D'Alia. Il testo della pregiudiziale QP2 spiega abbastanza bene perché voi abbiate deciso di utilizzare strumentalmente delle esigenze reali. reali. Nessuno di noi ignora infatti che esistono gogne mediatiche e circuiti perversi in cui cittadini che non c'entrano niente con i processi, ma anche gli stessi imputati vengono colpiti in maniera ingiusta e ingiustificabile, con la fuoriuscita di atti giudiziari coperti dal segreto istruttorio. dal segreto istruttorio. Tra l'altro, per rafforzare il diritto alla *privacy* con il presidente Marini e il collega Sanna abbiamo anche presentato una proposta mirata di riforma costituzionale per consentire una tutela maggiore. Tuttavia, utilizzare strumentalmente queste vicende per negare un funzionamento efficace dei processi con l'articolo 1, con l'astensione obbligatoria del giudice e la sostituzione del pubblico ministero, di cui hanno già parlato il relatore di minoranza Legnini e il collega D'Alia, previsione di tutta una serie di ostacoli per l'uso delle intercettazioni, a cominciare dalle autorizzazioni, significa negare l'equilibrio tra i diritti, che è il fondamento della Costituzione. Lo vorrei ricordare, in particolare, al collega Malan, che è un appassionato della Costituzione americana;

altri diritti goduti dai cittadini». Mi appello a questo emendamento che esprime il senso fondamentale del costituzionalismo moderno: l'idea dell'equilibrio tra i diritti. Voi, in nome di alcuni diritti che pure esistono nella nostra Carta e nella Carta di Nizza, ne sacrificate unilateralmente degli altri: è sacrificato il diritto dei cittadini alla sicurezza, rispetto al quale l'articolo 117 conferisce a questo Parlamento la legislazione esclusiva; colpite il diritto di cronaca e l'obbligatorietà dell'azione penale.

la definizione di Costituzione di un autore a lui caro: il generale De Gaulle. Diceva il generale De Gaulle: «Una Costituzione è un'ispirazione, delle istituzioni, una pratica». Ma per essere un'ispirazione ha bisogno di essere un punto di equilibrio tra le ispirazioni di tutti;

conterei di enunciare in rapida successione alcuni - non tutti, perché non sono ancora riuscito a trovarli tutti, in questo testo fittissimo di violazioni e di profili di contrasto con la Costituzione - i più macroscopici aspetti e profili di violazione della Carta costituzionale, per fare qualche brevissima riflessione, prima di sottoporre all'Aula la richiesta di non passare all'esame

scolastica - con la norma dell'articolo 21 della Costituzione. Il divieto di utilizzazione di intercettazioni legalmente disposte nella rigidissima griglia prevista dal testo che si vorrebbe approvare, laddove il reato venga derubricato, cozza contro l'articolo 112 della Costituzione, in materia di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale, e contro l'articolo 97 della Costituzione, in tema di efficacia, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione. La norma sull'astensione obbligatoria del giudice e la sostituzione del pubblico ministero vìola l'articolo 25 della Costituzione (norma peraltro recepita anche dagli atti sovranazionali in tema di giurisdizione), in materia di giudice naturale precostituito per legge. La norma in materia di sospensione cautelare automatica di giornalisti e altre categorie cozza contro l'articolo 27, comma secondo, della Costituzione, in tema di responsabilità personale. Le norme in materia di durata massima delle intercettazioni delle intercettazioni cozzano contro l'articolo 112 della Costituzione, in tema di obbligatorietà dell'azione penale, e generano quelle che con efficacia sono state indicate dal collega Legnini poco fa come indagini casuali e del tutto inefficaci. La norma in materia di guarentigia degli appartenenti ai servizi di sicurezza (ricordo che nella norma in questione si parla di mera riconducibilità delle utenze a soggetti appartenenti ai servizi) vìola l'articolo 3 della Costituzione, in tema di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. Le norme che equiparano le riprese visive non captative, le intercettazioni e le acquisizioni di tabulati, sottoposte in maniera incomprensibile (o forse troppo comprensibile) al medesimo regime, contrastano con il principio di ragionevolezza. Le norme che attribuiscono al collegio in sede distrettuale la competenza a disporre le intercettazioni (con quanto ne deriva in termini di spostamenti di carte, di dispendio di benzina, di energie lavorative, di ore uomo, di lesioni alla riservatezza e al segreto degli atti di indagine) cozzano con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione *ex* articolo 97 della Costituzione. Su questo punto lasciatemi dire qualcosa in più, per ricollegarmi a quanto detto poco fa dal collega D'Alia. La situazione che si viene a prospettare, se non fosse drammatica, se non fosse una campana a morto sull'efficacia delle indagini e sull'autonomia dell'attività investigativa e della giurisdizione, sarebbe grottesca. Infatti, un giudice singolo, il giudice per le indagini preliminari, continuerà ad adottare misure cautelari che durano a lungo e che restringono la libertà delle persone; un giudice singolo, in sede di giudizio abbreviato, avrà la facoltà di irrogare pene pesantissime, e un giudice distrettuale (tre uomini, tre donne, tre soggetti) dovrà invece decidere in tema di adozione o meno di un atto di ricerca della prova. Ciò è ridicolo o, meglio, sarebbe ridicolo e grottesco se non fosse tragico per il futuro, per l'efficacia per la sussistenza stessa delle indagini per una serie di gravissimi reati. Mi sia consentito di aprire e chiudere una parentesi. Non è vero che questa normativa non tocca le indagini in materia di criminalità organizzata e di terrorismo: le tocca da molti punti di vista. Le tocca perché i cosiddetti reati satellite diventano praticamente inindagabili con il mezzo delle intercettazioni e, quindi, al reato mafioso o al reato di terrorismo molto difficilmente si potrà giungere, così come oggi si fa, procedendo secondo una corretta sequenza investigativa. Ma vengono toccate quelle indagini anche per l'introduzione assurda di quella regola di giudizio per cui, per disporre un'intercettazione, è necessario adottare gli stessi criteri di giudizio previsti dall'articolo 192, commi 3 e 4, del codice di procedura penale. Questo ci porta ad un'ulteriore, clamorosa, violazione del principio di ragionevolezza. Davvero ho voluto fare questo *excursus* rapido, deliberatamente affannoso nel ritmo, per dare l'idea quasi fisica del senso di enorme disagio che noi tutti proviamo, che fuori da quest'Aula i cittadini provano rispetto ad un testo di legge che non tutela la riservatezza dei cittadini, ma la riservatezza dei criminali. il giorno prima (oggi) dell'adozione, che noi speriamo non si verifichi, di questa legge immaginiamo tre diverse categorie di soggetti: un gruppo di poliziotti, carabinieri, finanzieri che si riuniscono fra loro e sono in bilico tra la frustrazione, la rabbia e il senso di impotenza, perché non potranno continuare a fare il loro lavoro. Immaginiamoci un gruppo di giornalisti che si riuniscono fra loro e sono in bilico tra la rabbia, la frustrazione, l'impotenza di fronte alla tragica alternativa di essere ridotti al silenzio o di fare la difficile scelta della disobbedienza civile. Poi c'è un altro gruppo di persone: estortori, rapinatori, usurai, stupratori, corrotti, corruttori, ladri del denaro dei cittadini. Questi signori si accingono a brindare dandosi pacche sulle spalle. Da che parte stiamo? Da che parte sta la maggioranza? Chiedo di non passare all'esame del testo licenziato dalla Commissione.

ritengo che dall'esame del testo oggi all'ordine del giorno, anche da un esame non particolarmente approfondito, traspaia con tutta evidenza che il vero intento della maggioranza che l'ha concepito e che ora tenta di imporlo al Paese non è affatto quello di tutelare la *privacy*, bensì quello di limitare i poteri e i doveri investigativi della magistratura, la libertà di stampa e lo stesso controllo effettivo che il popolo dovrebbe essere messo in condizioni realmente di effettuare rispetto all'esercizio della funzione giudiziaria. Il popolo in questo caso non ha importanza: è molto più importante quando serve a giustificare eventuali provvedimenti di prepotenza. Il disegno di legge presenta diversi profili di illegittimità costituzionale e contrasta in più punti con diversi, sostanziali principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in particolare per quanto concerne i principi del corretto processo e della sua ragionevole durata, del diritto di difesa (articoli 24 e 111 della Costituzione, articolo 6 della Carta europea dei diritti dell'uomo, articolo 48 della Carta di Nizza), dell'obbligatorietà dell'azione penale (articolo 112 della Costituzione), nonché della stessa tutela della sicurezza (il diritto garantito in particolare dall'articolo 6 della Carta di Nizza). Mi soffermerò su aspetti che ritengo molto importanti e qualificanti (o dequalificanti) del disegno di legge in esame, equiparazione del regime di acquisizione dei dati di traffico a quello di ammissibilità delle intercettazioni. Questa norma, oltre a privare gli organi investigativi di un prezioso mezzo di prova, contrasta con il canone della ragionevolezza di cui all'articolo 3 della Costituzione, in quanto applica

Come evidenziato da una costante giurisprudenza costituzionale e di legittimità, infatti, la *data retention* concerne i soli dati esterni della comunicazione e non già, come invece le intercettazioni, il suo contenuto. La differenza a me sembra evidentissima. Né vale in proposito invocare la sentenza Malone della Corte europea dei diritti dell'uomo, che, pur ribadendo che «i verbali delle registrazioni contengono informazioni, in particolare soltanto ribadendo che «i verbali delle registrazioni contengono informazioni, in particolare soltanto i numeri chiamati, i quali costituiscono un elemento integrante della comunicazione telefonica» e che la consegna di queste informazioni alla polizia, senza il consenso dell'abbonato, si risolve in un'interferenza con il diritto garantito dall'articolo 8 della Carta europea dei diritti dell'uomo, non si è tuttavia pronunziata sull'opportunità di estendere a tali operazioni la disciplina delle intercettazioni. si consideri come tale nuova disciplina - ma questo forse non interessa alla maggioranza - comporterà invece un'indebita estensione dei tempi del procedimento, in quanto per la sola acquisizione dei tabulati sarà necessario addirittura il vaglio del tribunale collegiale

Non meno importanti sono gli effetti della normativa sul diritto di difesa: anche questo è stato evidenziato, ma vale la pena di rimarcarlo, perché la vittima in taluni

di disporre intercettazioni telefoniche, telematiche e soprattutto ambientali, possibili solo per reati distrettuali o permanenti, in virtù del requisito della necessaria finalizzazione all'osservazione dell'attività criminosa: ciò mi sembra a dir poco incomprensibile. si possa immaginare la predisposizione di intercettazioni ambientali per osservare l'attività criminosa, quando esiste nel nostro sistema l'obbligo preciso di intervenire nel corso della consumazione del reato per interrompere la consumazione dello stesso e quindi per evitare ulteriori gravi conseguenze. Generalmente, salvo rarissimi casi, non si interviene con l'intercettazione per osservare la consumazione di un reato, ma per acquisire fonti di prova indispensabili ad accertare la verità processuale e quindi ad assicurare i responsabili dei delitti alla giustizia: anche questo non sembra essere un problema della maggioranza. Acquisire tabulati, disporre videoriprese a contenuto captativo o in luoghi privati, prevedendo in particolare la competenza del giudice collegiale di un tribunale distrettuale, significa rallentare i tempi del processo e complicare gli stessi problemi in nome dei quali la maggioranza dice di essere partita nel nel formulare questo disegno di legge. C'è poi la sanzione dell'inutilizzabilità delle intercettazioni in altri procedimenti, qualora il fatto sia diversamente qualificato e per esso non ricorrano i presupposti per le intercettazioni.

cosa si fa, quando, invece che davanti alla cattiveria o alla "natura birichina" del pubblico ministero, ci troviamo davanti ad una derubricazione per effetto di fatti nuovi, di valutazioni fatte nel corso delle indagini e del processo, che successivamente inducono il giudice a valutare il fatto in maniera differente. pur non essendoci responsabilità alcuna di chicchessia, prenderemo i risultati delle intercettazioni telefoniche relative a reati per cui non è prevista l'utilizzazione dell'intercettazione e li getteremo nel cestino. Ciò, perché non serve accertare la verità, ma serve introdurre una serie di ostacoli per far sì che il giudice o il pubblico ministero ritardino o non siano in grado di accertare la verità dei fatti: questo è quello che traspare. I tempi del processo, inoltre, si allungheranno, e lo abbiamo già detto. Queste limitazioni, pur non applicandosi tutte ai reati distrettuali, avranno effetti deleteri - come è stato detto poc'anzi - anche sulle indagini relative ai cosiddetti delitti di mafia, in quanto non solo ostacoleranno significativamente l'attività investigativa relativa ai reati satellite o ai reati scopo dell'associazione, ma paralizzeranno l'attività dei tribunali distrettuali. Inoltre, neppure per i reati distrettuali si deroga alla previsione dei presupposti individualizzati per intercettare soggetti diversi da quelli indagati, che devono avere un collegamento diretto con le indagini o consentire un ricorso al parametro della colpevolezza. Anche questo - il rifarsi di procedura penale, che invece sono stati concepiti e scritti al fine dell'emissione di un provvedimento cautelare e non già di disporre un accertamento o un reperimento di fonti di prova evidente l'effetto limitativo di tali restrizioni sulle indagini, in particolare per i reati associativi o di concorso esterno in associazione mafiosa farà sgranare gli occhi a molti di voi!). Si consideri, inoltre, come le nuove ipotesi di astensione obbligatoria del giudice e del pubblico ministero per le dichiarazioni rilasciate sul procedimento, ovvero per la mera iscrizione del pubblico ministero nel registro degli indagati del reato, produrrà l'eliminazione o la messa al bando di quel magistrato. Ci si libera cioè del magistrato scomodo, violando quindi uno dei princìpi fondamentali della nostra Costituzione,

Il complessivo regime di pubblicazione degli atti procedimentali prevede il divieto di pubblicazione, e questo riguarda il diritto della stampa di esercitare un dovere: quello di far conoscere ai cittadini la verità su fatti che si stanno svolgendo all'interno della giurisdizione. eliminare il giornalista scomodo attraverso una semplice iscrizione nel registro degli indagati, e anche qui la presunzione di innocenza sembra non valere. Ritorna anche in questo caso il vecchio ritornello che bisogna colpire magistrati e giornalisti:

Infatti attraverso la competenza di un tribunale avremo un allungamento pericoloso e dannoso dei tempi ed un ampliamento della possibilità che vi possano essere fughe di notizie. Quindi, attraverso tale intervento emerge ancora una volta la prova che l'obiettivo dichiarato non è quello reale, perché ci sarà una maggiore possibilità che la *privacy* venga ad essere colpita. Per queste considerazioni chiedo che il provvedimento non venga preso in esame per manifesta contrarietà alle norme della nostra Costituzione.

credo che tutti noi, quando abbiamo sentito che si doveva trattare delle intercettazioni telefoniche, pensavamo di avere a che fare con la conciliazione di alcuni principi contenuti nella nostra Costituzione:

quindi, leggendo il testo di questo disegno di legge, che si sarebbe cercato di conciliare, meglio di quanto non l'avesse

sul deposito delle intercettazioni là dove si rendevano pubbliche immediatamente tutte le intercettazioni, perché si stabiliva l'obbligo di depositare tutti gli atti nei cinque giorni successivi al termine delle intercettazioni, a garanzia del diritto di difesa. Quindi tutte le intercettazioni venivano depositate: sia quelle che avevano una rilevanza ai fini del processo, sia quelle che riguardavano persone assolutamente estranee al processo. Ci aspettavamo anche che si cercasse di inserire la possibilità di pubblicare anche notizie che non attenessero strettamente al processo se avessero avuto una rilevanza notevole ai fini sociali. Di tutto si è parlato fuorché di questo; anzi, invece di soddisfare questi principi della nostra Costituzione, pare che invece si cominciasse proprio con il cercare di rendere addirittura impossibile il processo. Basti pensare all'articolo 1, commi 1 e 2, del disegno esame. Vorrei ricordarvi tali commi, poiché non hanno niente a che fare con le intercettazioni; essi hanno piuttosto a che fare con la possibilità di allungare i tempi del processo penale facilitando la criminalità, soprattutto quella organizzata, nell'esclusione dei giudici dal processo. si introduce un obbligo di astensione per il giudice se questi abbia pubblicamente rilasciato dichiarazioni concernenti il procedimento. Credo Credo che chiunque legga tale norma non possa non rendersi conto dell'irragionevolezza e quindi del contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, per il semplice fatto che è un'affermazione talmente generica generica e vaga che non si sa e non si capisce quali siano le dichiarazioni che obbligano il giudice ad astenersi dal processo.

Succede che il collegio deve essere cambiato. Se si tratta di un giudice monocratico, occorre far subentrare un altro giudice; se si tratta di un giudice collegiale, deve essere cambiato il collegio e, in tal modo, si deve ricominciare il processo dall'inizio. qualsiasi persona capisca quale rischio immenso corra un processo con una norma di questo tipo, che è assolutamente fuori da qualsiasi ragionevolezza. Ma c'è ancora di più, perché questo stesso principio si estende poi, nel comma 2, al pubblico ministero: anche il pubblico ministero che rilascia dichiarazioni, magari vaghe ed assolutamente

Questa è una delle seconde cause che allunga enormemente i tempi dei processi e quindi urta in maniera inequivoca, oltre oltre che con il principio di ragionevolezza di cui all'articolo 3, anche con il principio che abbiamo fissato nell'articolo 111, ossia con la ragionevole durata del processo.

che prevede la possibilità per il capo dell'ufficio di escludere dal processo il sostituto che se ne occupa nell'ipotesi in cui venga denunciato per rivelazione del segreto d'ufficio. Non c'è chi non veda che, a questo punto, specialmente nei processi di criminalità organizzata, si è fatto un grosso favore alla criminalità organizzata, che manderà ovviamente dei regali a chi questa norma voterà, perché basta fare una denuncia, anche infondata, nei confronti del magistrato scomodo perché questi possa essere escluso dal processo con un provvedimento del procuratore della Repubblica, sentito il

appartiene alla criminalità organizzata liberarsi di un pubblico ministero, magari nel punto cruciale del processo, facendo venir fuori una notizia riservata e ancora segreta e attribuendo il fatto al magistrato che dà fastidio.

sostituto (che magari ha un processo con 50 imputati, con indagini fatte con grande fatica e che conosce solo lui) e passare il procedimento a un altro sostituto che deve ricominciare tutto da capo.

che è stata iniziata e che viene portata avanti costantemente da quasi 20 anni. Credo peraltro che a nessuno sfugga che la delegittimazione di un'istituzione così importante

disegno di legge contrasta in maniera assoluta con la ragionevole durata del processo, di cui all'articolo 111 della Costituzione, è l'attribuzione al tribunale collegiale del distretto della decisione sulle intercettazioni telefoniche.

che può fare da solo, quando diventa GUP, in un processo di omicidio e dare l'ergastolo o 30 anni di reclusione per l'omicidio per cui è stato chiesto il rito abbreviato. fare attenzione, perché questa norma, una volta approvata, dovrà necessariamente comportare l'approvazione dell'altra disposizione che già fa parte del disegno di legge n. 1440 e che già è applicata in Campania e riguarda l'obbligo di emettere il mandato di cattura da parte del tribunale capoluogo del distretto, cui devono essere trasmessi tutti gli atti. Mi domando

decidono dell'80 per cento dei reati di criminalità organizzata, dovranno essere istituiti dei turni tra tutti i giudici per decidere sulle intercettazioni, sulle o le misure cautelari in generale. Tutti questi giudici diventeranno incompatibili a giudicare nel relativo processo;

Il senatore D'Ambrosio è al termine del suo intervento, ma ha il diritto di essere ascoltato da chi sta in Aula e credo sia dovere dei colleghi di ascoltare. D'AMBROSIO *(PD)*. Signor Presidente, le faccio notare che evidentemente la breve durata del processo interessa soltanto quando si intende introdurre un'altra causa di estinzione del reato; quindi, concludo qua il

«Pubblici siano i giudizi e pubbliche le prove del reato»: così ammoniva Beccaria, sottolineando come il segreto fosse il più forte scudo della tirannia. Ebbene, il nostro codice di procedura penale ha tradotto questo monito

comporta una trasparenza ed un'opportunità di conoscenza e di informazione, permettendo un effettivo controllo da parte dei cittadini. Si apprende come funziona la giustizia in generale e come evolvono i singoli casi giudiziari, i comportamenti e le capacità degli attori professionali del processo (giudici, pubblici ministeri ed avvocati). Tenere aperti i microfoni mantiene accesa l'attenzione ed impedisce insabbiamenti; consente a chiunque di farsi un'idea e, con quella, di schierarsi eventualmente tra innocentisti e colpevolisti; sentire le voci e, in alcuni casi, i volti dei protagonisti permette di percepire l'ambiente ed il clima sociale, culturale e politico I vantaggi sono evidenti: controllo dell'attività dei giudici e diffusione della conoscenza sul sistema legale nel suo funzionamento pratico. Fino a poco tempo fa, ritenevamo che il disegno di legge in materia di intercettazioni servisse fondamentalmente per cercare di tutelare la *privacy* dell'indagato, quello che ancora non è stato rinviato a giudizio; in questo testo, su cui richiamo l'attenzione - che, in realtà, interviene sulla pubblicità del dibattimento. mandato in onda (ed oggi mette a disposizione sul suo sito Internet) ben 15.599 udienze di processi, senza nessun taglio né selezione, nessuna mediazione giornalistica. È lo stesso modello adottato per le sedute del Parlamento; è una sorta di università popolare, è il conoscere per deliberare. Ora tutto questo è a rischio per l'incomprensibile norma che in un attimo chiuderebbe le porte delle aule giudiziarie, lasciando fuori proprio quel popolo italiano in nome del quale vengono emesse le sentenze. Signor Presidente, onorevoli senatori, abbiamo allegato nella questione sospensiva

che si sono potute registrare e dibattimenti che hanno avuto la possibilità di uscire dall'aula del processo e di arrivare agli ascoltatori di Radio Radicale;

devo dire che grande attenzione da parte di quella stampa che paventa il bavaglio non c'è stata. Mi auguro che se ne accorga, perché cancellare un pezzo della storia d'Italia, chiudere i microfoni dei processi sarebbe un atto sarebbe un atto di incomprensibile politica, che non avrebbe alcun senso: non si tutelerebbe l'indagato, non si tutelerebbe la giustizia, né l'imputato né il pubblico ministero né il giudice, nessuno. Non si capirebbe davvero la motivazione. *(Applausi

che viene oggi posta all'attenzione del Parlamento è di grande complessità e rilevanza. Si tratta di porre in rilievo l'applicazione e il rispetto di fondamentali princìpi costituzionali, a cominciare in prima analisi dall'articolo 15, il quale tutela la riservatezza delle comunicazioni personali. Anzi, l'ordinamento costituzionale prevede per questo diritto la tutela e la denominazione di diritti inviolabili ed impreteribili.

Ma vi è di più. Si tratta anche di giustapporre gli interessi fondamentali alla libera formazione dell'opinione pubblica e alla libertà di comunicazione e di espressione del pensiero, garantita e tutelata dall'articolo 21 della Costituzione. In tutto questo contesto credo sia sfuggito agli interventi dei colleghi dell'opposizione l'altro impreteribile contenuto dell'articolo 27, che è la presunzione di non colpevolezza,

la continenza dell'espressione e la rilevanza pubblica. Quante notizie sono state pubblicate sui nostri quotidiani che non rispondevano al canone fondamentale della verità! si tratta di introdurre un principio importante a tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, in un Paese in cui c'è un abuso delle intercettazioni telefoniche. è il Paese più intercettato, in cui la segretezza delle comunicazioni è la più limitata. La senatrice Poretti ha parlato poco fa di Cesare Beccaria; a me piacerebbe ripartire da Thomas Hobbes e da «Il Leviatano»,

probabilmente deve essere riscritta la pagina delle autonomie della polizia giudiziaria, del rapporto tra polizia giudiziaria e pubblico ministero, ma la norma che prevede - credo una garanzia effettiva, per cui la richiesta di intercettazioni deve essere sottoscritta dal sostituto, dal procuratore e dal giudice collegiale, non deve far venir meno questo principio di garanzia. Noi sottolineiamo il rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini e dell'attività della magistratura, ma pensiamo che gli abusi che in questo Paese sono stati commessi debbano venir meno. *(Applausi

favorire i momenti di confronto e di dibattito su un tema così delicato possa agevolare uno scambio di contatto, di idee tra maggioranza e opposizione. In questo senso i miei sforzi sono sempre stati finalizzati.

il ruolo di terzietà e di neutralità per essere garante dei diritti della maggioranza e dell'opposizione. In funzione del ruolo che ho cercato di svolgere su questo delicatissimo tema delle intercettazioni, cioè quello di

approccio in Commissione per poter riaffrontare alcuni temi contenuti negli emendamenti proposti dalla maggioranza che modificano il testo esitato dalla stessa Commissione possa costituire un elemento utile quale tentativo per trovare una sintesi di mediazione. Il mio tentativo è squisitamente finalizzato a questo compito e a questo obiettivo. Lungi da me dall'entrare nel merito delle valutazioni e delle proposte fatte dalla maggioranza e dei subemendamenti presentati dall'opposizione. Io rimango terzo nei loro confronti, ma ritengo che su questo tema il ruolo della Presidenza non possa e non debba sottrarsi dal favorire al massimo i momenti di confronto e di approfondimento che la stessa opposizione ha chiesto subito in Conferenza dei Capigruppo, una settimana orsono. In relazione a questo, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento, intendo rinviare alla Commissione giustizia i seguenti emendamenti, presentati dal senatore Gasparri ed altri, ed i relativi subemendamenti, presentati dall'opposizione: 1.700, 1.701, 1.702, 1.703, 1.704, 1.705, 1.706, 1.707, 1.708, 1.709 e 1.710. La Commissione giustizia dovrà pronunziarsi sui predetti emendamenti e relativi subemendamenti e riferire all'Assemblea a partire dalla seduta pomeridiana di martedì 8 giugno, alle ore 16,30.

*(PD)*. Signor Presidente, come tutti sapete, questa mattina all'alba un convoglio pacifista, diretto a Gaza per portare aiuti umanitari, è stato attaccato in acque internazionali da reparti militari dello Stato di Israele: 19 persone sono state uccise e molte decine ferite, di cui alcune gravemente. Si tratta di un fatto, come ciascuno può capire, molto grave; si tratta - questo almeno è il mio giudizio - di un'aggressione alla pace e alla stessa democrazia israeliana. Le conseguenze di questo fatto sono imprevedibili, ma sicuramente gravi per le reazioni che oggi abbiamo potuto ascoltare in tutte le parti del mondo. Penso, in particolare, alle reazioni europee, al fatto che molti Paesi hanno convocato gli ambasciatori dello dello Stato di Israele per avere chiarimenti e per esprimere la preoccupazione dei relativi Governi. Questa mattina, per fortuna, con una dichiarazione, il ministro Frattini ha corretto una prima dichiarazione del sottosegretario Mantica, che sembrava giustificare l'azione israeliana. Credo che correttamente si stia avanzando, da parte dell'Unione europea, la richiesta dell'apertura di un'inchiesta internazionale, garantita internazionalmente, che chiarisca le responsabilità e lo sviluppo degli avvenimenti. Ritengo, signor Presidente, che su una questione così grave sarebbe bene che il Ministro degli esteri riferisca in Parlamento sulla situazione e, naturalmente, sulle scelte che il Governo italiano intende fare. *(Applausi

Signor Presidente, ancora una volta richiamo l'attenzione sul problema della Phonemedia. In particolare, voglio sottolineare la situazione drammatica che già da tempo si è venuta a determinare per i suoi lavoratori e che tuttora non trova soluzione. Di recente l'azienda è stata commissariata e l'amministratore delegato indagato per bancarotta. Detto questo, i dipendenti non percepiscono lo stipendio dal mese di ottobre. Per cui, alla fine, sono stati gli unici a dover pagare concretamente, e con loro le rispettive famiglie. Il paradosso è che gli unici a pagare continuano ad essere i lavoratori, mentre i responsabili a tutti i livelli, compresi quelli che hanno concesso finanziamenti pubblici, non si attivano minimamente. Ora, è stata attivata la cassa integrazione, ma la burocrazia non si muove. Manca ancora la firma del Ministero dell'economia. A Novara molti parlamentari si erano attivati visto che sono componenti del Governo di centrodestra e della Lega Nord; ma poi non li abbiamo più visti e oggi i lavoratori sono tornati da noi, dall'opposizione, per chiedere aiuto.